La informo che il Presidente della Repubblica, con propri decreti in data odierna, adottati su mia proposta, ha accettato le dimissioni rassegnate dall'onorevole Andrea Ronchi dalla carica di Ministro senza portafoglio, nonché dall'onorevole Adolfo Urso, dall'onorevole Antonio Buonfiglio, dall'onorevole Roberto Menia e dal signor Giuseppe Maria Reina dalla carica di Sottosegretario di Stato, rispettivamente, allo Sviluppo economico, alle Politiche agricole, alimentari e forestali,

l'interno*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la problematica riguardante la sede del comando provinciale dei Vigili del fuoco di Ancona va inquadrata in un contesto più generale, che vede il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile fortemente impegnato in un progetto di rivisitazione, sotto il profilo logistico e strutturale, di tutti i comandi dislocati sul territorio nazionale. Il Dipartimento si propone, infatti, di assolvere al meglio la propria missione istituzionale a garanzia dell'incolumità dei cittadini, assicurando, nel contempo, la sicurezza degli stessi operatori del soccorso. L'attuale sede del comando provinciale dei Vigili del fuoco di Ancona, ubicata nel centro cittadino, è localizzata in un complesso di proprietà demaniale, costituito da quattro fabbricati. Uno di questi, di maggiori dimensioni, nonché realizzato di recente secondo moderni sistemi costruttivi (fine anni '90), rispetta i necessari standard in materia di sicurezza ed accoglie, ad oggi, gli uffici del comando provinciale e della direzione regionale dei Vigili del fuoco. L'attività di rimessaggio dei mezzi ed altra parte delle attività operative svolte dal comando sono state invece dislocate in *containers* o in sedi distaccate nell'ambito del territorio provinciale. Soltanto i due edifici meno recenti del complesso, realizzati alla fine degli anni '50, presentano condizioni di effettivo degrado. Infatti, gli stessi, più volte sottoposti a verifiche tecniche da parte di professionisti esterni incaricati dal Dipartimento, sono stati, di recente, dichiarati inagibili non più rispondenti alla normativa antisismica vigente in relazione alla loro epoca di costruzione. In tale contesto, certamente di particolare complessità, il Dipartimento, dopo aver valutato anche l'eventualità di una ristrutturazione e ricostruzione *in loco* dell'attuale complesso, d'intesa con la Direzione regionale ed il comando provinciale dei vigili del fuoco, ha avviato un percorso finalizzato alla individuazione di una sede alternativa, compatibile sotto il profilo economico, nonché idonea sul piano logistico e operativo ad accogliere gli uffici del comando. Tale percorso vede anche impegnate, come parti attive sul territorio, in un'ottica di leale collaborazione, il prefetto di Ancona, altri uffici periferici dello Stato e le stesse autorità locali. Sono attualmente in corso trattative con il Comune di Ancona per l'assegnazione di un'area da destinare alla realizzazione della nuova sede del comando provinciale dei Vigili del fuoco, individuata in zona stadio del Conero, e si confida di pervenire, in tempi ragionevolmente brevi, ad una soluzione definitiva. Nelle more dell'individuazione della sede ritenuta più idonea, il Dipartimento ha comunque adottato, anche attraverso l'erogazione delle opportune risorse, ogni misura necessaria a garantire le migliori condizioni di vivibilità e operatività dell'attuale sede della Direzione regionale e del comando provinciale dei Vigili del fuoco di Ancona.

Sono contenta del fatto che, comunque, si stia lavorando e spero in tempi brevi si trovi una area nuova per rispondere ad una esigenza importante del comando dei Vigili del fuoco.

non sarà attivato a pieno proprio per la mancanza di personale. Ricordo che non si è «uni e trini», almeno quando si fa i Vigili del fuoco, per cui sarà difficile che le medesime persone possano svolgere ovunque le stesse funzioni in modo opportuno

per l'interno*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le questioni sollevate nell'atto di sindacato ispettivo vanno inquadrate nel più ampio contesto delle diverse iniziative che, su molteplici versanti, sono state adottate proprio per garantire la migliore funzionalità degli uffici delle prefetture e delle questure Si tratta di misure imposte da esigenze di carattere temporaneo e straordinario, adottate per attuare specifiche strategie organizzative. La stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato, cui si riferisce l'interrogante, non è al momento consentita dalle esigenze di contenimento del disavanzo pubblico, che ha portato ad interventi di eccezionale rigore. Peraltro, le medesime esigenze di razionalizzazione e di contenimento dei costi delle pubbliche amministrazioni hanno imposto al Ministero dell'interno un'ulteriore riduzione delle dotazioni organiche del personale. D'altra parte, gli uffici di prefetture e questure fanno fronte ai relativi compiti d'istituto avvalendosi delle altre misure organizzative e di sistema che, a partire dal 2009, sono state adottate per la velocizzazione delle istruttorie e lo smaltimento dell'arretrato, facendo ricorso soprattutto sull'implementazione della tecnologica negli uffici. Sono state, infatti, assegnate agli uffici immigrazione delle questure 300 nuove postazioni di lavoro, anche al fine di consentire l'apertura di nuovi sportelli al pubblico. Sono state, altresì, distribuite 70 nuove apparecchiature *visascan* di ultima generazione, per il più rapido rilevamento delle impronte digitali. Si è provveduto, inoltre, ad affrontare situazioni di forte criticità degli uffici maggiormente impegnati, con l'invio *in loco* di un'apposita unità di intervento rapido, istituita presso la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere, una vera e propria *task force* specializzata per risolvere le problematiche via via emergenti. Le iniziative adottate hanno fatto registrare significativi risultati nella concessione dei titoli di primo soggiorno, nei rinnovi dei permessi e nei tempi medi di conclusione del procedimento.

con un incremento di oltre il 50 per cento. Dal 1° gennaio al 31 ottobre 2010 sono stati definiti con esito favorevole complessivamente 1.144.198 procedimenti relativi a titoli di soggiorno, comprendenti sia i rinnovi che i rilasci. Nello stesso arco temporale, sono stati emessi 4.022 provvedimenti di diniego. Si sono, inoltre, progressivamente ridotti i tempi medi assoluti di conclusione dei procedimenti: si è passati

Nel 2010, i tempi medi di produzione dei titoli di soggiorno risultano attestati intorno ai 40-45 giorni. Il *trend* di questi dati è suscettibile di progressivi, ulteriori miglioramenti, fino al raggiungimento dell'obiettivo dei venti giorni, previsto dalla legge, che il Governo intende perseguire. L'attività degli uffici, pertanto, non subirà né pause né soluzioni di continuità e ciò grazie all'implementazione delle tecnologie e alle misure organizzative adottate. Per quel che riguarda l'impiego di ulteriori 650 unità di personale, l'ordinanza di protezione civile n. 3828 del 27 novembre 2009 ha autorizzato il Ministero dell'interno e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali «ad utilizzare per un periodo non superiore a sei mesi, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestatori di lavoro con contratto a termine, nel limite massimo, rispettivamente, di 650 e 300 unità, da ripartire tra le sedi di servizio coinvolte nelle procedure di regolarizzazione del lavoro irregolare». Il ricorso a tale personale, per il quale si è provveduto alla copertura dei conseguenti oneri con le risorse derivanti dal versamento del contributo forfetario di 500 euro per ciascuna istanza di emersione dal lavoro irregolare, si è reso necessario al fine di consentire l'espletamento, in termini di urgenza, di tutte le misure organizzative indispensabili per una efficace gestione delle procedure amministrative connesse alle dichiarazioni di emersione. Il personale è stato infatti destinato esclusivamente all'espletamento dell'attività relativa alla procedura di emersione, con il risultato che ad oggi è stato evaso oltre l'80 per cento delle

che è in coerenza e in continuità con quella che ha dato al collega Minniti alla Camera. I dati che lei ha citato dimostrano un fatto inequivocabile: l'efficienza del lavoro di queste persone Queste persone di cui oggi lo Stato, il suo Ministero, vuole fare a meno. Penso che le esigenze non siano diminuite e non diminuiranno nei prossimi anni; e vi sono due livelli della questione posta, che intersecano quelli della politica. Il primo: vi è l'efficienza delle prefetture, del lavoro svolto da queste 650 persone vincitrici di un concorso sui temi dell'immigrazione, degli archivi, dei permessi di soggiorno, permettendo in questo modo alle forze di polizia di operare direttamente sulla strada per la sicurezza che tutti noi che facciamo politica invochiamo ogni giorno. Molti di loro hanno operato per 5, 6, 7 anni per le esigenze dello sportello unico; hanno accumulato esperienze e competenze che sarebbe assurdo perdere, sostituendoli - come lei ci ha testé comunicato, signor Sottosegretario Sottosegretario - con personale precario proveniente da cooperative, del tutto inesperto di queste difficili tematiche. Mi sembra un dato abbastanza discutibile. Vi è anche un secondo aspetto, meno appariscente ma che come esponenti della politica ci interroga maggiormente. Giustamente, è compito del Parlamento legiferare perché qualsiasi lavoratore non rimanga in stato di perenne precarizzazione presso aziende private. Le domando e domando a me stesso per il ruolo che occupo come parlamentare: è giusto che presso lo Stato, ovvero presso gli organi istituzionali periferici più rappresentativi dello Stato, le prefetture, alcune persone rimangano per cinque o per sette anni a svolgere con professionalità e competenza ruoli di responsabilità, senza prospettive e garanzie, e che oggi si comunichi in quest'Aula che non ci sono prospettive per queste lavoratrici e per questi lavoratori? Sono a chiedere al Governo un ripensamento ed una risposta più organica, dal momento che penso che le esigenze che lei ha evidenziato non verranno meno,

il Ministero dell'interno è particolarmente impegnato affinché le necessarie misure di contenimento della spesa pubblica degli ultimi anni non incidano negativamente sugli strumenti necessari al perseguimento della missione e dei compiti affidati dall'ordinamento al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Tra i principali versanti di impegno vi è proprio quello riguardante il contenimento al minimo della carenza di personale, pur nella impossibilità di coprire tutti i posti vacanti in organico. Infatti, sin dall'avvio della presente legislatura, in ragione delle elevate professionalità e dedizione degli operatori del Corpo, è stato avviato un percorso per assicurare un incremento delle risorse umane a garanzia del mantenimento

da ultimo la legge finanziaria per il 2010 che, per il triennio 2010-2012, prevede stanziamenti per assunzioni di personale del Corpo nazionale a copertura del 100 per cento Principio, quest'ultimo, confermato anche in sede di approvazione del più recente decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. Si tratta di interventi che, pur non essendo di per sé sufficienti ad azzerare l'attuale scopertura di organico del Corpo nazionale, potranno comunque consentire, al termine del triennio, un'inversione di tendenza rispetto al passato, fra personale collocato a riposo e e personale da assumere, tale da poter ragionevolmente prevedere una diminuzione delle carenze. In tale contesto generale si inseriscono le problematiche evidenziate dalla senatrice interrogante a proposito del personale del Corpo nazionale nelle Marche, con particolare riferimento al comando di Ancona, le cui carenze, pur consistenti, non rispecchiano i valori percentuali indicati nell'atto di sindacato ispettivo. Tali carenze, per il personale delle qualifiche operative (vigile, capo squadra, capo reparto), che rappresenta, numericamente, l'ossatura principale dei comandi sul territorio, si attestano al 16 per cento circa, in linea con altre analoghe realtà a livello nazionale. Si assicura, comunque, che verrà data la massima attenzione alle esigenze rappresentate dall'interrogante non appena sarà possibile procedere a nuove assegnazioni, sia a seguito della conclusione dei corsi di formazione semestrale per vigile permanente, avviati tra la fine del 2009 e l'inizio del 2010 nell'ambito delle assunzioni già autorizzate da disposizioni di legge; sia a completamento entro l'anno corrente delle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione di 814 vigili del fuoco; sia in sede di definizione delle procedure per i passaggi interni di qualifica (concorsi interni per caposquadra e caporeparto), attualmente in fase di svolgimento. Per quanto riguarda il parco automezzi, la relativa dotazione presso il comando di Ancona - che, attualmente, dispone tra i principali mezzi di soccorso di 4 autogru, 3 autoscale, 5 autobotti e 16 autopompe serbatoio - è in linea con lo standard nazionale. Peraltro, nonostante gli importanti sforzi già compiuti dal Governo con il primo provvedimento anticrisi, che nel contesto della drammatica emergenza sismica nella Regione Abruzzo ha assicurato al Corpo nazionale uno stanziamento pari a otto milioni di euro per la manutenzione, l'acquisto dei mezzi e la relativa gestione, la situazione complessiva dei mezzi operativi e, nello specifico, del comando di Ancona è certamente migliorabile. Al riguardo, si segnala che entro l'anno corrente è previsto un incremento del parco automezzi del Comando con l'assegnazione di due autopompe serbatoio e due autobotti. In merito alla situazione delle sedi di servizio del comando di Ancona e del distaccamento di Fano, si premette che il competente dipartimento del Ministero dell'interno, nella piena consapevolezza di dover assolvere al meglio alla propria missione istituzionale a garanzia dell'incolumità dei cittadini (assicurando, nel contempo, la sicurezza degli stessi operatori del soccorso), è fortemente impegnato, anche attraverso la destinazione di apposite risorse,

dopo aver valutato l'eventualità di una ristrutturazione e ricostruzione *in loco* dell'attuale complesso, è stato avviato un percorso per l'individuazione di una sede alternativa, compatibile sotto il profilo economico, nonché idonea sul piano logistico e operativo. Tale percorso vede impegnati, oltre alle strutture centrali e territoriali del dipartimento dei Vigili del fuoco, quali parti attive sul territorio, il prefetto di Ancona, le strutture periferiche dello Stato competenti in materia, nonché, in un'ottica di leale collaborazione, le stesse autorità locali. Sono attualmente in corso intese con il Comune di Ancona per l'assegnazione di un'area da destinare alla realizzazione della nuova sede del comando provinciale dei Vigili del fuoco, individuata in zona stadio del Conero, e si confida di pervenire in tempi ragionevolmente brevi ad una soluzione. Nel frattempo è stata, comunque, adottata ogni misura necessaria a garantire le migliori condizioni di vivibilità e operatività dell'unica struttura dell'attuale sede ancora agibile, ove sono ubicati gli uffici della direzione regionale e del comando provinciale dei Vigili del fuoco di Ancona. Per quanto riguarda il distaccamento permanente dei Vigili del fuoco di Fano, tenuto conto dell'inadeguatezza dell'attuale sede di servizio, è in atto il massimo impegno dell'amministrazione per assicurare agli uomini del distaccamento una nuova sede in grado di rispondere al meglio alle esigenze del soccorso tecnico urgente nel territorio interessato. È stata infatti già individuata un'area di proprietà comunale della superficie di 10.000 metri quadrati, da destinare alla realizzazione della nuova caserma dei Vigili del fuoco. Il percorso, volto a riaffermare il ruolo di centralità del Corpo nazionale fra gli apparati dello Stato preposti alla sicurezza nella sua più ampia accezione - che, come già anticipato in premessa, è stato avviato dal Governo nel corso della legislatura - trova riscontro anche sul piano dei riconoscimenti economici al personale. In particolare, sono stati adottati provvedimenti legislativi che, a partire dal riconoscimento del principio di specificità del ruolo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, al pari delle forze di polizia e delle Forze armate, contenuto nel primo provvedimento cosiddetto anticrisi adottato dal Governo e reso ancora più chiaro dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, in materia di lavori usuranti, hanno assicurato agli operatori del Corpo importanti passi in avanti sotto il profilo del trattamento economico. Con il richiamato provvedimento anticrisi il Governo ha inoltre stanziato risorse aggiuntive, da destinare in parte all'attuazione dei patti per il soccorso pubblico da stipularsi annualmente tra Governo e parti sindacali e, in parte, all'istituzione di una speciale indennità operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente espletato all'esterno. con decreto-legge n. 39 del 2009, cosiddetto decreto-legge Abruzzo, convertito dalla legge n. 77 del 2009, è stata ripristinata, a decorrere dall'anno 2009, analogamente a quanto già previsto per il personale dei comparti sicurezza e difesa, l'indennità di trasferta anche per il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Ed ancora, con il terzo decreto anticrisi, n. 78 del 2009, convertito dalla legge n. 102 del 2009, è stata autorizzata, a partire dal 2010, la spesa annua di 15 milioni di euro allo scopo di rifinanziare la speciale indennità operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente, istituita dal citato decreto-legge n. 185 del 2008. Si aggiunge, infine, che, in ragione della specificità del ruolo svolto è stata riconosciuta, con il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 126, anche al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco l'indennità di trasferimento, al pari degli altri Corpi dello Stato chiamati ad assicurare la sicurezza dei cittadini: indennità riconosciute da questo Governo che prima non erano riconosciute.

innanzitutto desidero ringraziare il Sottosegretario per la compiutezza della sua risposta e dichiarare la mia parziale soddisfazione,

chiaro allora che la soddisfazione rimane a metà. Resta invece del tutto positiva la sua ricognizione su quanto è stato fatto, anche come attenzione specifica ad un Corpo che ha la sua specificità

con tempestività e con un prudente e conseguente monitoraggio della questione, perché effettivamente le situazioni di sofferenza, dovute all'instabilità degli edifici e alla loro scarsa capacità di contenere contenere quanto deve esservi contenuto, rendono problematica la situazione. Dico di più: i mezzi che lei ha elencato

ricerca*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, su questa delicata vicenda, che si riferisce alla scuola romana di Sesto Miglio, la direzione generale dell'ufficio scolastico regionale del Lazio, sollecitata da questo Dicastero sui quesiti posti puntualmente dall'onorevole interrogante, oggetto del confronto odierno, ha prodotto una precisa e dettagliata relazione. La stessa cosa ha fatto il Ministero della salute, opportunamente sensibilizzato e chiamato a fornire gli elementi necessari a valutare il caso in questione, in quanto destinatario della medesima interrogazione. La direzione generale scolastica del Lazio riferisce infatti con nota n. 27266 dell'8 novembre, che il dirigente scolastico della scuola interessata, prontamente interpellato sul particolare avvenimento, ha comunicato che, accertata la diagnosi di tubercolosi polmonare nei confronti dell'insegnante, sono stati assunti immediatamente i dovuti contatti con il responsabile del servizio della medicina scolastica della ASL competente per territorio. Accertata la contagiosità del caso, lo stesso capo d'istituto si era preoccupato di avvisare tutti i genitori degli alunni delle due classi interessate e tutto il personale a più diretto contatto con la docente malata. I sanitari interpellati raccomandarono l'applicazione del protocollo sanitario, che prevede accertamenti progressivi mirati. Gli stessi inoltre precisarono che, per la malattia in questione, non fosse prevista alcuna forma di disinfezione né di chiusura temporanea della scuola. In quei giorni si procedette perciò, da parte del servizio di igiene e sanità pubblica della ASL di riferimento, all'applicazione puntuale di quanto previsto dal protocollo sanitario in caso di infezione tubercolare. Furono quindi ampiamente illustrate agli interessati le caratteristiche della malattia e del contagio e si resero note le procedure previste dal protocollo sanitario, comunicando a tutti i presenti le procedure già attuate e quelle programmate, impegnandosi verbalmente ad estendere gli accertamenti a tutta la popolazione scolastica del plesso e al personale secondo procedure e cadenze ben individuate. Venne, inoltre, sottolineato da parte del servizio di igiene e sanità pubblica della stessa ASL, che la trasmissione della tubercolosi avviene esclusivamente dal malato al sano attraverso l'aria, ed eventuali interventi di bonifica (sanificazione, disinfezione, sterilizzazione) ambientale non sarebbero stati effettuati, in quanto privi di qualsiasi efficacia pratica o preventiva. o preventiva. Ugualmente, in quella situazione, non avrebbe prodotto nessuna utilità, ai fini della tutela della salute, la chiusura delle scuole. L'ufficio scolastico regionale rimase comunque in costante contatto con il dirigente di Sesto Miglio, che ha continuato a mantenere sempre una stretta collaborazione con le strutture sanitarie coinvolte, agevolando il loro operato e tenendo sempre rapporti corretti e collaborativi con l'utenza ed il personale. C'è poi da osservare, partendo dai dati forniti a questo Ministero dal dipartimento della prevenzione e della comunicazione del Dicastero della salute, che l'attuale situazione epidemiologica della tubercolosi in Italia è caratterizzata da una bassa incidenza nella popolazione generale. Infatti il tasso grezzo annuale di incidenza della tubercolosi, sempre da quanto comunicato dal Ministero della salute, è in costante discesa: nel 2008 è stato pari a 7,66 casi per 100.000 abitanti. Ciò pone l'Italia al di sotto del limite che definisce la classificazione di Paese a bassa endemia (10 casi per 100.000 abitanti). Ai fini quindi della prevenzione della malattia tubercolare gli interventi più efficaci sono rappresentati dalla diagnosi tempestiva, dal trattamento efficace e dalla ricerca dei contatti dei casi, sia nei cittadini italiani che stranieri. Nessuna efficacia, come prima accennato, ha perciò la bonifica ambientale, peraltro non prevista dalle linee guida nazionali per il controllo della malattia. È necessario altresì sottolineare che anche dalla relazione dell'agenzia di sanità pubblica della regione Lazio, riguardante la stessa vicenda della scuola elementare di Sesto Miglio, cui si fa appunto riferimento nell'interrogazione in discussione, emerge, come già detto, che gli interventi opportuni di provata efficacia sono stati prontamente messi in atto dalle autorità competenti non appena avuta notizia del caso di tubercolosi, al fine di rintracciare tutti i contatti ed arginare il rischio di una possibile epidemia. In riferimento poi all'ipotesi di procedere con uno *screening* di massa, non ha alcun fondamento logico che gli accertamenti per la diagnosi di patologia tubercolare vengano effettuati di routine, ma esclusivamente nei nei casi in cui vi sia un sospetto su base clinica (per la sintomatologia presentata da un soggetto) o su base epidemiologica (per un possibile contatto con un caso accertato). Per quanto riguarda la diffusione della tubercolosi tra la popolazione immigrata, diversi accurati studi indicano come l'insorgenza della malattia si verifichi tra il primo e il secondo anno dell'arrivo in Italia, spesso a seguito del disagio sociale in cui vengono a trovarsi numerosi nostri immigrati. Come per la popolazione italiana, anche per gli immigrati gli interventi più efficaci sono rappresentati dalla diagnosi tempestiva, dal trattamento efficace e della ricerca dei contatti di casi. Anche per loro, quindi, c'è bisogno sicuramente di puntare su mirati interventi preventivi, svolti in collaborazione con le associazioni di volontariato e con i rappresentanti delle comunità, vigilando in modo particolare sui minori.

ringrazio il Sottosegretario per la risposta a questo atto di sindacato ispettivo, che porta la data del 19 maggio 2010. Faccio però notare al Sottosegretario che in questo atto ispettivo facevo richiamo anche ad un precedente atto di sindacato ispettivo presentato il 4 febbraio 2009, che faceva riferimento alla denuncia di casi di tubercolosi accertati nella scuola professionale «Don Minzoni» di Alghero (Sassari) e nella scuola professionale alberghiera di Senigallia (Ancona), di cui avevano dato ampia notizia gli organi di stampa. A questo atto ispettivo non è mai stata data nessuna risposta, quindi alcun seguito.

Credo però, signor Sottosegretario, che ci siano alcune questioni che dobbiamo affrontare. Se è vero che non è necessaria la bonifica ambientale perché non siamo in presenza di un fatto epidemiologico, come lei ha prima evidenziato,

che stanno caratterizzandosi soprattutto a livello infantile e nelle scuole e che interessano non solo gli alunni ma anche i docenti. Lei sa - e deve sapere, se non lo sa - che spessissimo, anche per deontologia professionale o per le leggi vigenti, nei certificati medici non viene definita la diagnosi. Quindi, ciò che io chiedo è che sia fatto nelle scuole un accertamento serio, invece: perché ora siamo in presenza di piccole zone, punte di un *iceberg* che probabilmente invece è molto più grosso. Se a voi non risulta, a me personalmente risultano diverse segnalazioni, dopo questi atti ispettivi che sono naturalmente diventati pubblici, di fenomeni di questo tipo. Come lei ben sa, naturalmente, è vero che non è l'ambiente in sé che può far insorgere la malattia, che si trasmette per via aerea e così via, ma se c'è una persona infetta lei sa meglio di me che proprio per questo, se questa persona infetta continua a frequentare ambienti particolarmente intensi dal punto di vista antropico, questa infezione si può naturalmente propagare. Io chiedo, e le chiedo, attraverso questo atto ispettivo, non solo di verificare i casi specifici e quindi anche quelli pregressi, rispetto ai quali non mi è stata data risposta, ma che questa benedetta medicina scolastica (parliamo sempre di prevenzione: la sanità parla di prevenzione, la pubblica istruzione si nutre anche di questo discorso preventivo che ha anche una valenza promozionale educativa sotto ogni profilo, perché la personalità riguarda anche la fisicità e la fisicità riguarda lo stato di salute *in primis*)

Depotenziato e quasi annullato questo servizio, non c'è più niente. Quindi, voi sapete soltanto quello che scoppia, che la stampa denuncia perché sono casi eclatanti. Sotto queste denunce c'è un mare di omertoso silenzio dovuto anche alle leggi vigenti che tutelano la *privacy*,

un'assunzione di responsabilità per un problema che oggi sembra piccolo o di facile soluzione, ma che un domani, considerata la multietnicità delle nostre scuole, la grande problematica sociale a cui andiamo incontro,

prevenzione e una programmazione seria, anche dal punto di vista della medicina scolastica, perché effettivamente questo servizio possa tornare ad essere espletato nella dimensione che aveva prima e con finalità ancora più aggiornate rispetto ai problemi e ai pericoli a cui